anche dal punto di vista dell'informazione pubblica. Signor Presidente, a breve lei darà comunicazione delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. visto, nella bacheca all'ingresso dell'Aula, che all'ordine del giorno vi è già il decreto-legge in materia di allontanamento dei cittadini comunitari, in cui viene specificato che il Presidente della Commissione riferirà

di avere necessità di intervenire nuovamente rispetto ai fatti che stanno accadendo, piuttosto elastici e flessibili, va bene, ma al limite della decenza.

Presidente, come già facemmo nel corso della prima lettura di questo provvedimento, noi socialisti esprimiamo su di esso un voto favorevole, sia pur accompagnato da molte perplessità. Il decreto indirizza ad aumento di spesa pubblica il maggior gettito emerso da giugno ad oggi, principalmente come risultato del recupero dell'evasione fiscale. Viene in tal modo indotto un peggioramento dell'indebitamento netto, pari a mezzo punto di PIL. Noi apprezziamo l'oggetto di questo decreto: il recupero dell'evasione, che ovviamente è uno dei punti più qualificanti. Di grande rilievo è anche il riconoscimento del principio di incapienza, che si concretizzerà in un rimborso monetario diretto a favore dei contribuenti a più basso reddito. Rintracciamo un'altra misura positiva: gli interventi sulle infrastrutture. Per quanto riguarda il resto, vediamo una totale assenza di interventi strutturali e una spesa che spesso si perde in mille rivoli improduttivi e insufficienti, perdendo così una grande occasione o per abbassare il debito pubblico e i relativi oneri finanziari, oppure per avviare politiche strutturali. A questo proposito, una delle aree importanti, direi indispensabili, delle politiche strutturali è quella dell'equità, cioè quella del*welfare*.

di legge finanziaria, su cui il nostro Gruppo, il Partito Socialista, aveva presentato un emendamento in tema di *welfare* che prevedeva un intelligente sostegno al reddito (subordinato alla sottoscrizione di un patto di servizio da parte dei lavoratori a progetto). Questo nostro emendamento fu ritenuto molto positivo dal Governo e dal relatore, tanto è vero che si tramutò in un ordine del giorno assai impegnativo, in cui si prevedeva che, per scelta di miglior contesto,

parlamentare: il rapporto, sia formale che fiduciario, fra il Governo e l'Assemblea. Per noi questa è una cosa assai grave, che da adesso in poi ci porterà a guardare sempre nel merito le questioni che il Governo proporrà, soprattutto mirando a due grandi aree di intervento: quella della crescita e della competitività e di politiche premiali per le imprese che investano per la crescita del Paese e quella per l'equità e la giustizia sociale. Quindi, nell'annunciare questo «voto perplesso» favorevole a questo provvedimento (per i motivi di contenuto che ho appena detto), annuncio che il nostro voto favorevole sul decreto del *welfare* a valle dell'inganno che il Governo ha perpetrato in Aula avverrà solamente perché l'Esecutivo, come si sa, porrà la questione di fiducia. Signor Presidente, colleghi, torna all'esame di quest'Aula per l'approvazione definitiva il decreto fiscale collegato alla finanziaria, contenente fondamentali misure volte al perseguimento di importanti obiettivi per lo sviluppo e l'equità sociale Come è noto, il testo in oggetto è il frutto di un percorso operoso intrapreso dalle due Camere; un percorso approfondito nel quale si è inteso modificare il testo originario del Governo, con l'intento di rendere il più possibile efficaci le disposizioni in esso contenute. Si tratta di disposizioni rivolte in particolare ad una platea che ricomprende fasce deboli della popolazione, come gli incapienti, per i quali è stata prevista una detrazione fiscale, quale rimborso per il 2007, pari a 150 euro. L'importo è stato correttamente rimodulato alla Camera per innegabili esigenze di copertura non soddisfatte, con l'impegno del Governo a riportare il *bonus* a 300 euro nel 2008. i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio delle abitazioni, con particolare attenzione alle giovani coppie con la predisposizione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica che valorizzerà il patrimonio demaniale, mettendo a disposizione un cospicuo numero di alloggi. i soggetti danneggiati da trasfusioni infette e per i talassemici. Altre importanti misure di politica sociale sono contenute nel provvedimento, come il piano straordinario dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'aumento delle risorse del 5 per mille, l'incremento del fondo per le politiche sociali e, ancora, le risorse per l'obbligo d'istruzione. Il decreto, che contiene dunque molte scelte positive ed equilibrate, opera un dedicato bilanciamento tra esigenze di risanamento e di ridistribuzione delle risorse e necessita quindi, di sollecita approvazione, considerando la sua imminente scadenza. Per queste ragioni, a nome dei Popolari-Udeur, confermo il giudizio ampiamente positivo sul provvedimento in oggetto, dichiarando pertanto il voto favorevole del Gruppo UDEUR.

perché si debba dare al Ministro la possibilità di ridiscutere un accordo raggiunto dopo lunghe discussioni con tutti i Comuni interessati in presenza di non si sa quali novità, visto che tale evento risale a cinque anni fa. Il terzo è relativo all'articolo 26, che riguarda le produzioni energetiche rinnovabili. Non siamo d'accordo che si debba continuare ad affrontare le questioni attraverso regali e regalie a progetti economici, a investimenti e a investitori volta per volta. Occorre un piano energetico nazionale; se ne sono dotati gli altri Paesi e non si comprende perché non debba farlo l'Italia.

sarà un inverno freddo e che siamo alla carretta. C'è bisogno di un minimo di serietà sui conti e sulle scelte reali che si vanno a fare. Ma vi è di più: un errore che secondo noi va recuperato, che dà

come ci accade da un po' di tempo a questa parte - voteremo a favore del decreto perché complessivamente ci sono altri punti positivi. Non potendo votare articolo per articolo, dando un giudizio generale, dichiariamo il nostro voto a favore. Perdo un istante per soffermarmi sulle questioni ideali che hanno spinto il senatore Dini a porre delle questioni sulle conquiste, sulle impostazioni, sulle rivendicazioni delle parti sociali più deboli del Paese. Egli ha posto grandi questioni ideali sulle quali dovrei soffermarmi a lungo, trattandosi di questioni ideali - e quest'Aula ha tanto bisogno di respirare alto - importanti per il nostro Paese; trattandosi delle questioni ideali del senatore Dini, ho già finito.

Ricordo che per la prima volta dal 2002 in quest'Aula riusciamo ad adottare provvedimenti che riguardano la finanziaria senza apposizione del voto di fiducia. voto di fiducia. Sottolineo che nell'Aula più difficile, quella del Senato dove i numeri sono quelli che tutti conoscono, siamo stati capaci di fare un discussione franca, serena, serrata, a volte anche di forte contrapposizione, ma in ultimo abbiamo votato senza il ricorso alla fiducia. Rammento a me stesso che in altri tempi, anche recenti (negli ultimi tre anni, per la verità, della passata legislatura), con numeri ben più forti e sostenuti di quelli che oggi sorreggono l'attuale maggioranza, in quest'Aula fu necessario ricorrere alla fiducia. Oggi tutto ciò è stato possibile perché, ad onta di quel che si legge ogni tanto, c'è una forte convinzione del ruolo del Parlamento da parte di questa maggioranza. Siamo una coalizione articolata e complessa - come sono solito ripetere - ma che ha nella centralità del Parlamento il suo punto di riferimento: quindi, discussioni, ma poi capacità di decisione sulla base sulla base di provvedimenti analiticamente esaminati e sui quali si trova larga condivisione. Credo che la manovra finanziaria si caratterizzi quest'anno (il decreto fiscale ne è la prova più evidente, ma il discorso vale più

extragettito, di possibilità di interventi non previsti nel programma perché probabilmente da un anno e mezzo o da due anni a questa parte i cittadini italiani hanno avuto la consapevolezza e la certezza che questa maggioranza e questo Governo non tollerano più zone franche,

questa maggioranza ha già indicato alla Nazione, ai cittadini italiani come intenderà usare il prossimo extragettito, che è facilmente prevedibile anche per il 2008. Abbiamo già detto con chiarezza che, dopo aver dato alle imprese (penso al cuneo fiscale e alla riduzione dell'IRES e dell'IRAP che realizziamo con questa manovra), sia venuto il momento di restituire e redistribuire ai cittadini virtuosi. Ritengo che questa maggioranza debba continuare ad insistere su tale strada con un no fermo all'evasione fiscale e debba cominciare una redistribuzione verso altri settori che finora potrebbero sembrare maltrattati rispetto alla redistribuzione in atto. Sequesta maggioranza farà ciò, continuerà ad esistere e a vivere bene. Per quanto ci riguarda, noi dell'Italia dei Valori controlleremo che ciò sia fatto.

Desidero semplicemente ribadire il giudizio sostanzialmente positivo dei senatori e delle senatrici del Gruppo della Sinistra Democratica,

modifiche che hanno migliorato il testo iniziale. Ne ricordo solo alcune: le misure in materia di gestione dei servizi idrici, gli interventi correttivi in materia di editoria, di enti locali,

modificato sostanzialmente il provvedimento; ha introdotto alcune modifiche positive; ha corretto un emendamento che era stato approvato in Aula al Senato, sul cui contenuto siamo d'accordo ma per il modo come era stato votato e per la copertura che era stata individuata, non poteva non essere corretto. Ricordo anche che nel corso della discussione in quest'Aula abbiamo approvato l'emendamento sugli emotrasfusi, che rappresenta uno dei due interventi - questo e quello contenuto nel disegno di legge finanziaria - che riesce finalmente ad affrontare una questione che si trascinava da tantissimo tempo.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, oggi va in scena il terzo tempo del secondo atto di quella commedia degli equivoci che si chiama Governo Prodi. Prodi. Siamo al terzo tempo del secondo atto bastava recarsi in qualunque luogo di riunione del Paese (un treno, un aereo, una sala d'aspetto, una riunione sindacale o politica, uno luogo d'incontro) per constatare che nessuno degli elettori italiani dichiarava di avere votato per la maggioranza e per il Governo che ne era scaturito. Questo non riscontrare nessun orgoglio del risultato elettorale da parte degli elettori era il classico segno dello scollamento totale tra un Governo e l'intero elettorato.

ben un anno, ha portato la maggioranza, e in particolare i principali partiti di questa maggioranza, a compiere un atto mai visto in un Paese democratico, cioè la sostituzione del *leader* prima di aver perso le elezioni, atteggiandosi e sentendosi come se si fossero perse le elezioni. Non esiste altro modo, infatti, di interpretare la decisione di procedere alla nascita del Partito Democratico e di incoronarne *leader* qualcun altro rispetto al capo del Governo, che ne dovrebbe essere l'espressione. È esattamente questo che si fa quando, perdendo le elezioni, si ritiene il pro*prio leader* non più all'altezza.

L'assurdità è che tutti i colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto, anche quelli che non hanno parlato oggi in quest'Aula, hanno sistematicamente preso le distanze dal Governo e dal gesto che stanno annunciando di compiere, cioè dal voto favorevole. Non ho ancora sentito in quest'Aula, e dubito che sentirò, un annuncio di voto favorevole convinto in favore del Governo. Se leggiamo quello che scrive sui giornali il collega Dini, riconosciamo in lui un fiero esponente di opposizione alla politica del Governo e non certo qualcuno che sarà qui a dare un voto favorevole. L'articolo pubblicato l'altro giorno sul «Corriere della Sera» era esemplare per la capacità di penetrante critica della strategia complessiva di politica economica, di cui questo decreto è un pezzo. Eppure il voto del collega Dini e di quanti a lui si riferiscono arriverà puntuale. Se poi leggiamo le dichiarazioni di ieri di Rifondazione Comunista in ordine ad un altro pezzo molto importante della strategia economica del Governo, cioè il Protocollo sul *welfare* e la decisione del Governo di apporvi la fiducia, troviamo un altro esempio di critica penetrante contro il Governo, ma dalla parte opposta, che si traduce in quest'Aula nuovamente in un voto favorevole.

Quindi, in realtà il risultato netto di tutte queste parole è che il Governo si mantiene in piedi a dispetto di se stesso e a dispetto del Paese. allora chiedersi, in termini di scienza della politica, come tutto questo sia possibile, perché tutto ciò accada. Vede, Presidente, il punto cruciale è che questo sarebbe un bel gioco, se la politica fosse corpo separato rispetto al Paese e variabile indipendente rispetto alla vita dei cittadini. Ma così non è. Il risultato è che le tensioni politiche di questa maggioranza, che si scaricano attraverso il diverso modo di configurarsi dei provvedimenti di politica economica, fanno sì che tali provvedimenti siano volti ad un solo fine, la sopravvivenza dell'Esecutivo,

la sua *constituency* elettorale, i suoi elettori. Abbiamo un Governo che fa accettare in Commissione alcune misure di cambiamento e poi le revoca quando decide

potere. Quando il potere si allontana dalla sua legittimazione democratica (e ciò è avvenuto in modo clamoroso lo scorso anno, quando si è determinata una distanza tra il Paese reale e il Governo, tanto che i partiti di maggioranza si sono sentiti in dovere di ristrutturarsi e di darsi un nuovo *leader*,

è stato realizzato solo al fine di garantire la sopravvivenza di chi è oggi al potere, a dispetto di chi si pretende di rappresentare.

Non capisco come si possa da parte della sinistra, dopo aver chiesto ed imposto che in un programma elettorale ci fossero alcune decisioni su quella che chiamano la precarietà del lavoro, sulla legge Biagi e sulla riforma previdenziale, vedersi da un voto di fiducia annullate tutte le proprie istanze, quelle per le quali - mi consenta, Presidente - ha lottato per cinque anni (per tre della legislatura (per tre della legislatura in cui quelle misure furono approvate e per due di questa). Un voto di fiducia fa cancellare la loro stessa esistenza. Colleghi, abbiate tutti quanti un minimo di sussulto di dignità. Guardate in faccia la gente che avete e state ingannando. Ciascuno di voi, ciascuna delle forze che disconosce in quest'Aula e disconoscerà sempre di più il Governo,

il Senato si accinge a licenziare in terza e definitiva stesura il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008. L'obiettivo perseguito da questo Governo e con tale decreto, così come fu anche con il decreto-legge dello scorso luglio (entrambi non per caso chiamati "tesoretto"), è di restituire e redistribuire risorse al Paese, specialmente alle fasce più deboli. Nella valutazione del provvedimento in esame, infatti, non si può non ricordare che la prima finanziaria varata da questo Esecutivo è stata prima di tutto una finanziaria del rigore, la quale ha perseguito soprattutto l'obiettivo del risanamento, visto e considerato che il bilancio dello Stato era gravato da un pesante debito pubblico ereditato da decenni del passato. Purtroppo, l'obiettivo perseguito con la scorsa finanziaria è stato molto poco e mal comunicato al Paese, con la conseguenza che i sacrifici che sono stati chiesti ai cittadini e alle imprese non sono stati capiti ma subiti come delle ingiustizie. Condividiamo, dunque, la scelta adottata ora dal Governo di utilizzare le risorse aggiuntive a disposizione e provenienti dall'extragettito soprattutto per la redistribuzione e lo sviluppo. È infatti giusto e doveroso che dei frutti di una politica economica rigorosa possano usufruire quei cittadini e quelle imprese che, con il loro sacrificio, hanno contribuito al risanamento, sopportando un aumento della pressione fiscale. Accogliamo - ribadisco Accogliamo - ribadisco - l'aver scelto la redistribuzione, ma chiediamo allo stesso tempo al Governo di non dimenticare che lo spazio di manovra è molto ridotto e che il Paese non può assolutamente permettersi un aumento della spesa corrente, la quale comporterebbe altre ed ulteriori tasse. Non penso solo ai rigidi paletti, quali i vincoli europei; penso soprattutto - e non mi stancherò di ripeterlo e di ripeterlo ancora - al debito pubblico e ai suoi interessi. Il fardello che l'Italia si porta dietro ormai da vari anni è di oltre 1.600 miliardi di debito, il più alto dei Paesi europei, che ogni anno costano allo Stato, ossia a noi tutti, una cifra di oltre 70 miliardi di interessi passivi. Quanto più pesante resterà questo fardello, tanto più difficile resterà coniugare il risanamento dei conti pubblici con concrete misure di impulso allo sviluppo, di riduzione della pressione fiscale e con interventi per ridurre le disuguaglianze sociali. Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento perché ritiene che, specialmente al Senato in prima lettura, sia stato compiuto un buon lavoro, sia in Commissione che in Aula. che al Senato, anche in prima lettura, il testo è stato approvato senza voto di fiducia. Entrando nel merito del provvedimento, accogliamo con favore che il decreto interviene a favore dei cosiddetti incapienti, ossia a favore di quelle persone che non possono mai beneficiare delle detrazioni fiscali perché il loro reddito è talmente basso che non possono pagare le tasse. Accogliamo con favore anche le misure agevolative sulle fonti rinnovabili,

nello specifico a sostegno della maternità e delle donne lavoratrici con bambini. Bisogna, infatti, rendere compatibile il lavoro delle donne, spesso indispensabile per la sopravvivenza della famiglia, con

con tutti i problemi e i risvolti conseguenti di sostenibilità del sistema pensionistico, sociale in generale, della sanità e dei casi di non autosufficienza. Al riguardo presenteremo a breve un disegno di legge e chiedo fin d'ora, sia alla maggioranza che all'opposizione, di sostenere questo obiettivo affinché tornino ad aumentare le nascite anche in questo Paese.

Oltre a ciò, incentiviamo l'obiettivo di rafforzare le strutture ferroviarie per favorire il trasferimento del traffico merci e delle persone dalla gomma alla rotaia. Al tempo stesso*,* però, ci troviamo d'accordo con le dichiarazioni rilasciate recentemente dal Ministro delle infrastrutture, onorevole Di Pietro, che non intende più concedere risorse al buio. Pur con il sostegno fornito in questi anni, le Ferrovie continuano ad annunciare nuovi rincari dei biglietti. Occorre pertanto trasparenza su dove finiscono questi soldi e, soprattutto, devono essere visibili ai cittadini viaggiatori e alle imprese i frutti di questi finanziamenti.

non sono sfruttate e, se lo sono, sono sfruttate molto male. Chiediamo dunque con insistenza che le Ferrovie utilizzino questi finanziamenti per migliorare le strutture e i servizi, allo stato assai carenti, e per porre rimedio alle indecenti condizioni igieniche nei vagoni dei treni. Concludo, signor Presidente, annunciando che il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al provvedimento in esame, con la richiesta, tuttavia, di perseguire sempre lo scopo di raggiungere un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di risanamento, una più equa distribuzione della ricchezza, soprattutto con riferimento alle categorie più deboli ed alle famiglie, e una riduzione del peso fiscale anche per le imprese.

migliorano la copertura finanziaria di alcune norme sulle quali c'era dubbia coerenza costituzionale.

alla modifica del Patto di stabilità al fine di non dover rinunciare ai fondi comunitari che necessitano di un cofinanziamento.

noi come altra parte del nostro schieramento siamo portatori, trovassero alcune prime risposte. Ricordo

che ha destinato una parte delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e

va vista anche collegata alle altre misure che abbiamo assunto all'interno della finanziaria, che caratterizzano in maniera più marcata una scelta di inizio di un percorso di redistribuzione sociale, soprattutto nei confronti dei cittadini pensionati, dei lavoratori meno abbienti e delle famiglie; una politica di maggiore equità, anche qui una politica che tenta di ricostruire, sotto alcuni aspetti, un minimo di Stato sociale dopo gli arretramenti e le demolizioni

un minimo di inversione di tendenza e di giustizia sociale nei confronti dei meno abbienti e dei cittadini italiani, a partire dai pensionati, dai giovani e dai lavoratori che si trovano in queste condizioni.

vivere una precarietà che è determinata non solo dall'incertezza del futuro del lavoro, ma soprattutto dall'impossibilità di programmarsi la vita perché le condizioni salariali sono quelle che

dovute alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale - che va ulteriormente incentivata -, penso che queste dovranno essere in primo luogo utilizzate per

ed alcuni nostri amici dell'opposizione, che la soluzione della questione salariale nel nostro Paese si risolva

perché attraverso la continua riduzione del costo del lavoro abbiamo sostanzialmente disincentivato le nostre aziende ad intervenire e ad investire sulla ricerca e sull'innovazione che sono gli unici elementi che danno competitività.

Si era lavorato all'interno della maggioranza e in un confronto stretto con il Governo per trovare soluzioni, dopodiché sono bastati i ricatti della Confindustria e di alcuni parlamentari, che purtroppo sono determinanti, per far sì che quel provvedimento sofferto - che non risolve i problemi dei lavoratori sia relativamente alle pensioni sia relativamente alla questione della precarietà

che il nostro continuerà ad essere un voto convinto se questa maggioranza, ed il rapporto tra l'Esecutivo e la sua maggioranza, continuerà ad essere quello che abbiamo verificato nel corso dell'esame di questo provvedimento di legge e della discussione sulla finanziaria.

delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi» viene concessa "una detrazione fiscale", quella di cui tanto si è discusso.

dice: che bello, ci saranno ancora dei tesoretti, finalmente potremo intervenire nei confronti delle categorie che hanno sempre pagato le tasse e che stanno soffrendo di un carico fiscale così pesante,

del *bonus*, della detrazione fiscale per gli incapienti, potrà essere ripristinato nel 2008, con le risorse là reperite, magari nell'ammontare che il Senato, nella lettura precedente di questo decreto, aveva indicato in 300 euro.

il ripristino di altri livelli per gli importi per gli incapienti. Nel momento in cui, invece, diciture di questo tipo vengono poste a livello legislativo, ciò vuol dire che neanche a livello politico ci si fida di quello su cui ci si accorda all'interno della maggioranza.

inqualificabile, all'interno di un disegno di legge. In attesa di un qualcosa che verrà, intanto facciamo questo, a livello legislativo. Ebbene, si tratta di un evidente segno dell'incongruenza e dei non accordi all'interno della maggioranza che ci sono ormai su tutto,

una situazione, quindi, che continua ad essere assolutamente precaria. Di precario, colleghi, non ci sono solo i lavoratori: c'è anche una maggioranza di Governo che in questo modo non riesce a dare le risposte che vorrebbe dare a livello programmatico, e delle enunciazioni del Ministro dell'economia (e che i cittadini si aspettano), di risanamento del debito pubblico,

La produzione industriale continua in maniera altalenante. Non vi è quindi una crescita della produzione industriale che permetta di sostenere anche lontanamente tutto l'intervento che, a livello di assistenzialismo e di spesa pubblica, la maggioranza di centro-sinistra sta mettendo in atto quotidianamente, decreto dopo decreto, finanziaria dopo finanziaria.

del rigore, del controllo della spesa pubblica e del debito pubblico, del controllo della pubblica amministrazione. Ricordate cosa era scritto nel vostro programma a proposito del fenomeno della burocrazia nel nostro Paese, della burocrazia che occlude spazi, impedisce la crescita e lo sviluppo di imprese e quindi di vero lavoro. L'unico lavoro che riuscite a pensare di creare è quello derivante dalla trasformazione dei precari in lavoratori stabili, ritenendo che sia un modo di generare un lavoro vero e concreto, che dia risposte occupazionali al Paese, quando sapete benissimo che così non è.

la patrimonializzazione delle imprese, il costo che, nell'insieme, la macchina pubblica ha nei confronti del complesso dello Stato e quindi il grave fenomeno, che dura da tantissimi anni, del drenaggio di enormi risorse della parte sana e produttiva del Paese a favore della parte improduttiva e anche poco sana. Perseguite queste strade perché in questa direzione volete

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questa legge di conversione del decreto-legge 159 si lega alla conversione del decreto‑legge n. 81 del luglio scorso, alla finanziaria alla finanziaria per il 2007 e a quella per il 2008, in corso di discussione alla Camera. Perché c'è questo collegamento?

da qualche mese. Queste maggiori entrate derivano però da un aumento della pressione fiscale. Nel 2007, è stato ricordato più volte e da più parti,

Il secondo motivo è il maggior gettito fiscale, che, secondo la Corte dei conti, si dovrebbe attestare nel 2007 intorno a 18-19 miliardi Queste maggiori entrate hanno costituito ben due tesoretti, che sono stati spartiti dall'attuale maggioranza con uno scambio di voti, in particolar modo al Senato, per tenere uniti i diversi dissidenti e i vari pezzi della maggioranza, soprattutto quelli più recalcitranti.

resto dei 18 miliardi e mezzo di maggiori entrate andrà ad alimentare la finanziaria. Come sono state utilizzate queste maggiori entrate? Bisogna tener conto di un punto fermo in questa discussione: l'articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007. Tale comma era chiaro, anche perché, meno l'UDC, fu approvato sia dal centro-sinistra, sia da una parte del centro-destra.

qualora nel corso dell'esercizio finanziario fossero state realizzate maggiori entrate da tributi, queste dovevano essere destinate prioritariamente

le rispettive leggi di conversione, che hanno ovviamente ampliato la platea dei beneficiari delle spese ivi previste, ci rendiamo conto che solo i cosiddetti incapienti, ossia coloro che non hanno reddito (ovvero hanno un reddito così basso che non pagano le imposte), avevano diritto prioritario alla restituzione fiscale. Quindi, tutti gli altri beneficiati

un impegno politico del centro-sinistra quindi maturato all'interno della maggioranza, avrebbe anche potuto coinvolgere il consenso di una parte del centro‑destra. Infatti, mentre i redditi medio-bassi hanno goduto di detrazioni e deduzioni fiscali, solo coloro che non pagano le tasse non hanno potuto godere di alcunché e non parlo degli evasori, ovviamente, ma di coloro che non raggiungono la soglia del minimo di imposizione fiscale (siano lavoratori autonomi, dipendenti o addirittura nullatenenti), tanto da meritare la cosiddetta imposta negativa, che sarebbe quella che riguarda gli incapienti, ossia il pagamento da parte dello Stato di un valore di imposta pari ai benefici che avrebbero ottenuto se avessero potuto pagare le tasse perché percettori di reddito.

che lo Stato restituiva anche ai senza reddito o percettori di basso reddito, come ho detto. In quella occasione, dove la maggioranza fu battuta in quest'Aula, si discusse sulla bontà della copertura finanziaria, ma non sul merito, sulla validità della scelta fatta. Si ritenne da parte di tutti che si trattava di un *fiscal drag* per i poveri, in linea con la norma e l'impegno politico del comma 4, come ho ricordato, della finanziaria 2007. 2007. Tale scelta era già stata fatta - è vero - dal Governo, che proponeva 150 euro, ma veniva rafforzata da un voto dell'opposizione che raddoppiava l'importo da 150 a 300 euro e quindi era una misura di grande significato sociale, di grande giustizia sociale.

rinunciare alle misure clientelari ed elettoralistiche contenute nel decreto, destinando le risorse alla riduzione del debito pubblico e noi avremmo quindi di una sfida virtuosa, non di una sfida in qualche modo diretta a limitare l'azione della maggioranza, ma a limitare quell'azione rivolta soltanto a soddisfare gli interessi di parte. Noi anteponevamo gli interessi del Paese a quelli della vostra parte. Invece, non solo avete conservato le misure che aumentano la spesa corrente e il disavanzo rispetto a quello che si sarebbe registrato a legislazione vigente, aumentando il fabbisogno e il debito pubblico che pagheranno le future generazioni, ma avete anche privilegiato la spesa corrente inutile e improduttiva a danno di quella sociale e agli investimenti per lo sviluppo. Questa, come ricordava il collega Stracquadanio, è la vera è la vera bollatura che viene fatta in senso negativo da questo Governo e da questa maggioranza. Questa è la peggiore pratica di Governo che si possa conoscere nella storia

nessuno lo ha dimostrato, né in quest'Aula né in Commissione né in altra sede: nemmeno il Ministro dell'economia e delle finanze, con la relazione prevista dal comma 5 della finanziaria 2007, che lo impegnava a dimostrare la natura e la tipologia di queste entrate.

e non si destina un euro per lo sviluppo, quindi abbiamo una pressione fiscale che si somma a risorse che non vengono date allo sviluppo.

vicenda politica dell'utilizzo dell'extragettito, o avremmo fatto un uso virtuoso di queste risorse? Sono convinto che se avessimo avuto un'Aula con un altro sistema elettorale, con soggetti politici derivanti da quest'altro modello, saremmo stati tutti più liberi di fare gli interessi del Paese anziché quelli di una sola parte. Ecco allora che la vicenda

Signor Presidente, colleghi senatori, l'*iter* parlamentare del provvedimento in esame mi induce a richiamare una nostra proposta di riforma del Senato (illustrata in un convegno del nostro Gruppo di alcuni mesi fa e presieduto dal vice presidente Caprili, con la partecipazione di altri esponenti di quest'Aula di maggioranza e di opposizione), maggioranza e di opposizione), tesa ad affermare la persistenza di una doppia lettura dei provvedimenti legati alla sessione di bilancio, anche in una ipotesi di Senato delle Regioni ad elezione diretta, non certo quel pasticcio votato alla Camera. Mi riferisco alla norma di cui all'articolo 44 del decreto in esame inerente le misure a favore dei contribuenti a basso reddito, di cui molti colleghi hanno parlato, il cosiddetto *bonus* incapienti, dove alla Camera si è corretta una copertura sbagliata, basata sull'attivazione del 30 per cento dei fondi dormienti che non sono attivabili, come ben sappiamo, avendo lavorato sul loro utilizzo anche in finanziaria in direzione della stabilizzazione dei precari. Vorrei allora soffermarmi su una specificazione sia politica, che tecnica.

al di là di qualche facile battuta, si è anche introdotto il principio di una misura fiscale permanente a favore dei contribuenti a reddito più basso, a quei soggetti passivi di imposta in attesa dell'introduzione - si afferma nel testo - di una disciplina organica, "di una misura fiscale volta ad assicurare il riconoscimento di una imposta negativa per i soggetti a basso reddito". Non è ancora il reddito sociale di cittadinanza che vorremmo, misura di *welfare*, ma è un primo passo, almeno sul terreno fiscale, per dare un segnale di risarcimento sociale ai soggetti più deboli. Un secondo aspetto riguardo la natura di questo intervento - lo ha ricordato su un altro terreno il collega Ciccanti - è la riduzione della pressione fiscale, il richiamato articolo 1, comma 4, della finanziaria

sul tema generale dell'extragettito, oltre che sulle misure specifiche: da una parte, l'extragettito per diminuire la pressione fiscale a partire dai più deboli, come avviene in gran parte, o, per altri versi, per ridurre il *deficit*, come pure con questo provvedimento avviene, in piccola parte, riducendo il saldo netto da finanziare. Una delle due ipotesi è sbagliata, non possono essere entrambe giuste. Allora, in contraddizione con entrambe le ipotesi, sento che

in netto contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, l'uno basato sulla questione della Tabella C,l'altro sui fondi discrezionali, insomma senza una copertura realmente sensata per una forza di governo.

sul lavoro dipendente. Allora, ecco il punto: con il decreto-legge abbiamo avviato una strada che va sicuramente potenziata. E basta con le polemiche sulla spesa corrente sempre improduttiva! Pensiamo alle ferrovie; per mesi avete detto che erano fermi i cantieri. C'è uno stanziamento in relazione alle ferrovie e francamente ci preoccupiamo più che il ministro Di Pietro fermi questo trasferimento perché vuole rendere i binari aperti ai privati, piuttosto che del fatto che quel tipo di stanziamenti può essere utile a rilanciare una fase di ripresa economica. Sugli altri punti del decreto, per brevità, non mi soffermo, perché hanno già detto e bene i colleghi Albonetti e Martone richiamando il piano di edilizia pubblica, i programmi di cooperazione internazionale, gli asili nido ed altri temi, primo fra tutti la moratoria per gli affidamenti ai privati del servizio idrico integrato. Quello su cui voglio soffermarmi è un punto politico. Su questo provvedimento, e più in generale legge finanziaria, abbiamo lavorato molto e bene in Commissione bilancio e in Aula nel Senato della Repubblica, con l'unità dialettica della maggioranza, senza ricorrere al voto di fiducia.

della sua maggioranza che vota un testo sul quale il Governo non pone la fiducia ma la mette su un altro. Qualcuno nella maggioranza già prima ha parlato di unità solo sul merito, da adesso in poi. Il nostro Gruppo condivide molto le parole del Presidente della Camera sul *vulnus* democratico di un voto di fiducia non sul testo approvato in Commissione. Al Senato questo non è avvenuto finora e credo che non avverrà. Il nostro Gruppo è preoccupato anche di posizioni che, in nome della concertazione con le parti sociali, rifiutino un confronto in ossequio ai *diktat* della Confindustria. Nel merito è importante parlare sempre, ma serve una finalità condivisa, serve coniugare rigore, equità e sviluppo, applicando il programma dell'Unione. Votiamo senza avverbi, non - come qualcuno ha detto - con convinzione, con meno convinzione o altro. Votiamo a favore del decreto-legge perché, oltre che sul merito specifico, ci ritroviamo sulle finalità generali del collegato e della manovra finanziaria. Il Partito della Rifondazione Comunista e la sinistra sono forze serie, radicate nel Paese, e devono guardare a grandi interessi sociali e popolari. Speriamo - mi rivolgo al Governo - di poter continuare a dire la stessa cosa anche per altri provvedimenti. Dipende dalla capacità dei movimenti di permeare l'agenda politica del Governo stesso, dal senso di responsabilità del Presidente del Consiglio e dei signori Ministri, e anche da alcuni settori della maggioranza, parafrasando il principe napoletano De Curtis, meglio noto come Totò - vorrei ricordare che ogni pazienza ha un limite. *(AN)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei motivare tre motivazioni sulla base delle quali il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre La prima motivazione è nel titolo stesso del decreto. Il collega Tecce ha giustamente ricordato Totò, che ogni pazienza ha un limite, ma ogni limite ha la sua pazienza. Vorrei rovesciare questa condizione, perché il titolo del provvedimento supera ogni limite di decenza, più che di pazienza. È È un decreto-legge recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria», e fin qui d'accordo; segue: «per lo sviluppo e l'equità sociale».

dei famosi 41 centesimi al giorno per gli incapienti. Quanto alla seconda motivazione, il decreto è tornato dalla Camera

Signor Presidente, così come è stato modificato dalla Camera, questo decreto mi ha ricordato molto un vecchio cartello appeso nella macelleria della piazza del mio paese tanti anni fa.

«oggi si fa credito, domani no». Infatti, si consente alle amministrazioni di sforare nel 2007 a condizione di una promessa di rientro nel 2008,

La seconda modifica consiste nella cosiddetta correzione del *bonus* per gli incapienti. Si è detto che l'emendamento Rossi, che raddoppiava da 150 a 300 euro l'*una tantum*

Se è un problema di copertura, dopo aver speso 7 miliardi e mezzo con il decreto di luglio e 8 miliardi e mezzo con questo decreto, per un totale di 16 miliardi, voi della maggioranza, che a parole fate maggior riferimento alle istanze sociali, dovreste spiegare perché

concedere 81 centesimi al giorno agli incapienti ponete un problema di copertura che tecnicamente non esisterebbe; infatti, un parallelo un parallelo contenimento in Tabella C avrebbe dato la copertura necessaria. La terza motivazione è la più grave, siamo di fronte ad un'operazione che somiglia alla legge del contrappasso. L'anno scorso il Governo aveva clamorosamente sbagliato tutte le previsioni di finanza pubblica.

di maggiori tasse e di maggiori spese. Nel corso di quest'anno, ha fatto emergere il falso in bilancio, chiamato tesoretto, e si è illuso di poter spendere quel di più di gettito che sta spendendo in questo momento:

nell'illusione - al rovescio, rispetto all'anno scorso - che le condizioni di crescita economica e di finanza pubblica, nella prospettiva 2008, potessero reggere questa operazione.

scenario economico europeo ed internazionale per fare quattro calcoli e constatare che le risorse che adesso state distribuendo non ci sono più? State distribuendo risorse in *deficit spending*, perché è automatico l'effetto sulla crescita dell'anno prossimo, che non sarà dell'1,5 per cento, ma sarà abbondantemente sotto l'1

non c'è sviluppo, non c'è redistribuzione sociale del reddito e c'è la prospettiva di una pericolosa emergenza finanziaria, che voi state costruendo in questi giorni, con questi vostri provvedimenti, aumentando di 24 miliardi

un'immagine che mi viene in mente e che non avrei mai voluto citare in quest'Aula. Nel mio paese, un vicino paese di campagna, nei favolosi anni Sessanta, un saggio sindaco dell'allora Partito Comunista tentò in Consiglio comunale di spiegare ai suoi assessori e ai suoi consiglieri la situazione difficile della sua amministrazione comunale, dicendo: cari colleghi, cari assessori, guardate che quest'anno abbiamo la prospettiva di un *deficit* dirompente, insostenibile per il nostro piccolo Comune. E allora l'altro saggio assessore dell'allora Partito Comunista, che aveva un nomignolo molto simpatico (si chiamava "il Cucco", qualche collega riconoscerà in questo il paese di Chiaravalle, nelle Marche), si alzò in piedi e disse: caro sindaco, ma se la situazione è così tragica e abbiamo tutto questo *deficit*, ebbene, spendiamoci pure quello! È ciò che questo Governo e questa maggioranza stanno facendo. *(Applausi

è notizia di pochi giorni fa che il reddito *pro capite* spagnolo ha superato quello italiano. Ma qualcuno nel Governo si è chiesto il perché di questo? Ci si è chiesti se leggi come quella che sarà posta in voto fra poco ci avvicinano alla crescita del PIL spagnolo o fanno crescere il reddito degli italiani come quello degli spagnoli - mi limito alla Spagna e non ad altri Paesi europei concorrenti più diretti - o se invece per caso ce ne stanno allontanando? Ci siamo chiesti se strumenti come quello che stiamo esaminando ci spingono all'ineluttabile o se sia il caso invece di fare qualcosa per cambiare una strada che sembra accettata e segnata senza nessun anelito di cambiamento? Ha senso - l'ha detto recentemente un illustre collega riprendendo motivi che erano stati sollevati da questa parte politica proprio in quest'Aula - procedere in un meccanismo di «*spend as you go*», che poi è inevitabilmente seguito da un meccanismo di «*tax as you spend*», cioè di crescita illimitata della spesa pubblica? Ha senso proseguire in questa strada? Ha senso approvare un decreto-legge che non ha altra funzione che quella di redistribuire in qualche modo, finanziando il collateralismo politico, il cosiddetto tesoretto che si era accumulato? Ma se di tesoretto si tratta, bisogna porsi almeno tre domande, signor Presidente.

accanto a queste misure, si stiano realizzando quelle riforme strutturali che ci potrebbero mettere nelle condizioni di resistere sui risultati acquisiti, o se invece se invece ciò non sia vero e viceversa si stiano realizzando delle controriforme vere e proprie che ci porteranno poi a perdere anche quel poco di buono che è stato fatto nel passato. È sotto gli occhi di tutti quanto sta avvenendo con questo decreto‑legge, ma ancora di più con una legge finanziaria e con un provvedimento sul *welfare* che stanno distruggendo giorno dopo giorno quei piccoli mattoni di credibilità che si erano andati costruendo in questo Paese. Allora veniamo alla prima domanda: esiste un tesoretto? Il gettito è cresciuto? Il gettito continua a crescere? È ragionevole pensare che sia mantenuto anche nell'ultima parte di quest'anno? Secondo me, signor Presidente, non è ragionevole, per una diversa quantità di incognite. La prima incognita è che l'aumento della tassazione imposta a partire dal decreto-legge del luglio dell'anno scorso ha causato e continua a causare seri problemi alle imprese italiane, vedono assottigliarsi sempre di più i margini di profitto proprio in un momento nel quale invece è necessario ricostituire i profitti per affrontare con possibilità di successo la sfida internazionale. È sotto gli occhi di tutti l'andamento del PIL. Molte imprese, molti amici imprenditori in questa fase vedono paurosamente muti i fax e i telefoni perché, dopo l'andamento soddisfacente che si è avuto fino a qualche mese fa, si inizia ad intravedere un tunnel oscuro. Il valore

spiace dirlo - la politica della Banca centrale europea continua ad essere di stretta monetaria e quindi non agevola la ripresa dei Paesi europei in un momento in cui l'inflazione è un rischio, ma forse non quello peggiore. A fianco di questi motivi di preoccupazione si unisce quello gravissimo della crescita del prezzo del petrolio, crescita che motivi geopolitici inducono a ritenere non passeggera ma duratura e forse destinata a consolidarsi nel tempo. Le famiglie italiane sono passate da un meccanismo di ampio risparmio ad uno di credito al consumo sempre più elevato, con la difficoltà ad arrivare a fine mese. La crescita delle esportazioni è solo in valore e non in quantità, e quindi riflette i maggiori costi che ha il nostro sistema Paese. È il momento di alleggerire detti costi. Rispetto a questo non si fa nulla, anzi si aggravano le condizioni della finanza pubblica; si aumenta la tassazione; non si agevolano, malgrado le parole che si sono sentite in occasione della legge finanziaria,

in ogni caso, la spesa non è di per sé buona. È una visione della sinistra quella di ritenere che comunque la spesa pubblica sia un bene. A mio avviso, non è così. Comunque, è un bene la spesa privata, è un bene lo sviluppo, è un bene lo sviluppo, ma ogni euro in più di spesa pubblica prima o poi inevitabilmente finirà per riflettersi in un euro in più di tassazione, anche se cerchiamo di dilazionare il problema,

per il risparmio e per gli investimenti delle imprese. Ogni euro in più di spesa non fa altro che rendere più gravi e pregiudicare le possibilità di sviluppo per il futuro del nostro Paese. Paese. Infine, signor Presidente, non possiamo nasconderci che qualunque risultato di tipo contingente di finanza pubblica, per essere mantenuto, necessita delle indispensabili riforme strutturali che allontanino i rischi incombenti che l'Italia ha, come molti Paesi europei, ma anche più di essi. Rispetto a questo dato, nulla si fa, anzi, si fanno consistenti e pericolosi passi indietro rispetto al passato. L'esempio della legislazione in tema pensionistico è solo la punta dell'*iceberg* di quello che sta avvenendo. Una controriforma *in peius* dei meccanismi pensionistici, tale che per salvaguardare qualche anziano prepensionando pregiudica gravemente i diritti e le speranze soprattutto dei giovani, condannandoli, questo sì, ad un mondo di vita precaria e di scarse prospettive, è la peggiore eredità che il Governo potrà lasciare al futuro ed alle prossime generazioni. Non è, però, solo una questione di pensioni; è anche una questione di prospettive del lavoro. La controriforma della legge Biagi significa

di Sinistra nel congresso del 1997: è meglio lavorare anche in modo precario piuttosto che non lavorare. Invece voi state spingendo

Si è addirittura proceduto ad una controriforma del sistema dell'istruzione che ci porta indietro, come se potessimo vivere ancora in un mondo dai confini chiusi quando invece è indispensabile far sì che i nostri giovani siano più propensi ad affrontare ad armi pari rispetto ai loro concorrenti internazionali il mondo dell'impresa e del lavoro. non sembra interessare. Come non sembra interessare - e torniamo ancora una volta al cuore del problema - un meccanismo nel quale la spesa pubblica viene considerata come uno strumento per oliare il consenso sociale. Quindi, l'unico effetto è quello di avere un consenso temporaneo a danno ancora una volta delle prospettive delle generazioni future, perché, come mi sono permesso di dire prima, la spesa pubblica sarà inevitabilmente seguita da un incremento della tassazione. E un incremento della tassazione perseguito - l'abbiamo visto in molti casi - a volte più con finalità punitive che non con finalità di sviluppo del reddito dei cittadini e delle potenzialità delle imprese è uno strumento gravissimo che penalizza un sistema che deve lottare con forza contro la concorrenza internazionale in questo difficilissimo momento. Per questi motivi, signor Presidente, credo che l'assalto all'arma bianca che viene fatto con questo decreto e con il disegno di legge finanziaria ai soldi, ai sudati risparmi ed alle tasse degli italiani sia la dimostrazione più evidente che questo Governo non ha la capacità di voltare pagina, di impostare una politica anche culturalmente diversa; non ha altro desiderio che quello di arrendersi ad una sorta di ineluttabile declino. Questo non può essere consentito, prima di tutto nelle nostre menti e nel nostro cuore e dopo nel nostro portafoglio. Credo, in conclusione, sia giunto proprio il momento di aprire le finestre e fare entrare aria nuova nella finanza e nella politica italiana.

Il decreto-legge n. 159 che l'Aula si appresta a convertire in legge si colloca solo apparentemente nel solco della tradizione che si è affermata nelle ultime sessioni di bilancio, a partire dalla scorsa legislatura. Una tradizione che vedeva accompagnare la presentazione alle Camere del disegno di legge finanziaria unitamente all'adozione di provvedimenti di decretazione d'urgenza tecnicamente collegati alla manovra di bilancio, orientati al perseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario fissati dalla stessa manovra. II decreto-legge n. 159 segna in tal senso una discontinuità di assoluto rilievo politico. Infatti, è la prima volta che un decreto-legge collegato alla manovra di bilancio, invece di concorrere alla correzione dei tendenziali, assume un carattere espansivo, distribuendo risorse mirate al rilancio degli investimenti infrastrutturali e al sostegno alle fasce sociali più deboli, impegnando somme pari a circa 8 miliardi e mezzo di euro. Un primo segnale in questo senso si era già avuto con il decreto n. 81 del luglio scorso, con il quale venne effettuata un'operazione di redistribuzione dell'extragettito fiscale pari a 0,4 punti di PIL, in quel caso orientata in prevalenza a sostenere i redditi dei pensionati al minimo e dei giovani con redditi discontinui. Quello distribuito con il decreto-legge n. 159 è dunque il secondo extragettito del 2007; sommato al precedente, porta a circa 15 miliardi di euro l'importo complessivo delle manovre espansive realizzate dall'inizio dell'anno da questo Governo e da questa maggioranza. A rendere possibile questa operazione eccezionale è stata una *performance* dei conti pubblici per il 2007 largamente migliore delle attese, riconducibile soprattutto al successo delle politiche di *tax compliance* messe in atto dal Governo fin dall'inizio della legislatura. Tutto ciò ha consentito in corso d'anno non solo di recuperare risorse aggiuntive da destinare allo sviluppo e all'equità sociale, ma anche di rispettare e per certi versi perfino di accelerare il programma di riduzione dell'indebitamento concordato in sede comunitaria. Ma soprattutto, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo fin dall'approvazione della scorsa finanziaria e con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il DPEF 2008-2011, con il decreto n. 159 viene avviato finalmente quel processo di restituzione del maggior gettito fiscale da tempo atteso dai cittadini, dando priorità a un intervento straordinario di sostegno ai soggetti economicamente più deboli che rimane senza precedenti per la sua portata - checché ne dica il senatore Baldassarri anche dopo il ripristino alla Camera dell'importo originariamente stabilito per il cosiddetto *bonus* imposto dalla manifesta insussistenza della copertura finanziaria dell'emendamento che lo aveva strumentalmente innalzato, e non certo del proponente. In particolare, alle famiglie con redditi così bassi cui non competerà il pagamento di imposte e che dunque non possono pienamente accedere alle agevolazioni fiscali riconosciute alle altre famiglie di lavoratori e pensionati, si riconosce un *bonus* straordinario di 150 euro per ciascun componente, secondo il modello dell'imposta negativa, adottato con successo in altri Paesi, a partire dalla Germania. Si tratta di un intervento nel segno dell'equità fiscale, significativo anche ai fini del sostegno allo sviluppo, specialmente nell'attuale congiuntura di rallentamento della crescita. Esso consente, infatti, di immettere nel sistema economico circa 2 miliardi di euro attraverso i maggiori consumi delle famiglie interessate dalla misura, con ciò concorrendo a sostenere la domanda interna e in particolare i consumi delle famiglie, oggi segnalati in flessione. Di analogo segno sociale deve ritenersi anche il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con il quale vengono destinati a tal fine 550 milioni di euro per far fronte all'emergenza abitativa nei Comuni insieme ad altri 150 milioni per la creazione di una società di scopo partecipata dall'Agenzia del demanio, con l'obiettivo di realizzare 80.000 nuovi alloggi entro dieci anni. Queste disposizioni, unite al pacchetto di interventi fiscali sulla casa previsto dalla legge finanziaria, costituiscono il primo nucleo di quel piano casa con il quale il Governo intende rispondere ad una delle più drammatiche emergenze sociali che affliggono storicamente le città, in particolare i grandi centri urbani, cioè la crisi degli alloggi. Coerentemente questa maggioranza ha ritenuto di riservare al problema della casa, nell'ambito della manovra finanziaria 2008, la parte più rilevante dell'investimento sociale per un importo complessivo pari a circa 3 miliardi di euro. Se la manovra correttiva realizzata nel luglio 2006 si connotava soprattutto per la sua portata redistributiva, il provvedimento attuale si caratterizza anche per la forte spinta agli investimenti in infrastrutture viarie su tutto il territorio nazionale. Ad essi sono, infatti, destinati 3,4 miliardi di euro comprensivi sia dei finanziamenti ad ANAS ed FS per il completamento di opere stradali e ferroviarie già cantierate, sia delle nuove risorse destinate all'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, allo sviluppo della rete metropolitana nei tre grandi conglomerati urbani di Roma, Milano e Napoli. Ammodernare, potenziare le infrastrutture del Paese, recuperare al Mezzogiorno l'economia produttiva sono fra i presupposti fondamentali affinché il nostro sistema economico possa colmare il ritardo di competitività e di crescita rispetto ai principali Paesi europei. Con questa manovra finanziaria questo Governo e questa maggioranza confermano il proprio impegno a voler dotare il Paese di una rete di infrastrutture al passo con i tempi. A testimoniarlo il fatto che essa destina alle infrastrutture un importo complessivo pari a quasi 35 miliardi di euro. Alle risorse stanziate dal decreto si aggiungono, infatti, i 7 miliardi di euro complessivamente stanziati dalla legge finanziaria per il rifinanziamento delle opere previste dalla legge obiettivo per il triennio 2008 2010. risorse che, a loro volta, si aggiungono agli oltre 3 miliardi di euro già destinati a tal fine dalla precedente legge finanziaria per l'anno 2008. Tale dato è tanto più significativo in quanto la media annuale degli investimenti infrastrutturali registrata nella precedente legislatura é stata appena di 1,8 miliardi di euro. Un anno fa, signor Presidente, onorevoli senatori, in questa Aula il Ministro dell'economia e delle finanze presentava i risultati della *due diligence* compiuta sulla situazione economica e finanziaria del Paese. Il Ministro ci consegnava allora dati oggettivi che ci riproponevano in termini molto obiettivi ciò che sentivamo essere fonte di forte criticità per il Paese. In primo luogo, vi era il gigantesco debito pubblico (il più alto in Europa e il terzo al mondo in valore assoluto): 1.600 miliardi di euro - visto che le statistiche piacciono ad alcuni colleghi - che ci obbligano a reperire ogni anno 70 miliardi per il pagamento dei relativi interessi; 1.200 euro all'anno in media, senatore Baldassarri, a testa, per ogni italiano, compresi i neonati. In secondo luogo, emergeva l'ampiezza dell'evasione fiscale, anch'essa del tutto fuori linea rispetto alla media europea con un divario che ammonta a 5-6 punti di PIL (75-90 miliardi di euro per ogni anno). Un anno dopo, in un tempo relativamente breve, siamo tornati in questa Aula a discutere della manovra finanziaria per il 2008 con una situazione sostanzialmente e profondamente diversa da quella dello scorso anno. Oggi ci è consentito raccogliere frutti della precedente manovra che è stata certamente dura, ma che presentava una missione chiara degli obiettivi da conseguire che oggi - possiamo affermarlo - risultano conseguiti. La nostra crescita economica è superiore alle stime, sono migliorate le entrate tributarie, la spesa è in linea con le previsioni. Anche al di là di ogni valutazione politica di merito, ad attestare il cambiamento di passo della gestione dei conti pubblici sono i dati che indicano una riduzione del*deficit* pubblico al 2,4 per cento, l'incremento dell'avanzo primario dallo 0,1 al 2,6 per cento, la flessione del debito pubblico dal 105 al 103 In conclusione, signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico-L'Ulivo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159, del 2007, esprimiamo l'auspicio che la strategia di ripresa della crescita economica, messa in atto dal Governo fin dall'inizio della legislatura, possa dispiegarsi pienamente in linea con gli obiettivi congiunti di risanamento dei conti pubblici, di recupero di efficienza e di produttività del sistema economico, di sostegno sia delle categorie più povere della popolazione, sia delle situazioni più disagiate all'interno del Paese, a cominciare dal Mezzogiorno. Signor Presidente, gli argomenti utilizzati dalla destra per denigrare ciò che non è criticabile non hanno nulla a che vedere con l'impostazione liberale che loro propugnano perché strizzano l'occhio solo al peggiore populismo di facciata. Il risanamento, lo sviluppo, l'equità sono queste i tre obiettivi e i tre valori reciprocamente connessi e non necessariamente interdipendenti che si confermano gli obiettivi guida delle politiche economiche e sociali del Governo di questa legislatura.